consentire agli operatori una più corretta interpretazione del loro modo di agire nel trattamento delle acque reflue, in maniera tale da non incorrere in eventuali complicazioni interpretative da parte degli

inquinamenti dovuti ad acque reflue o a scarichi di tipo industriale o a scarichi in mare, che tanto danno stanno recando e di cui tanto abbiamo parlato nei mesi scorsi. Abbiamo voluto inasprire le pene per dare uno strumento ancora più inflessibile nella valutazione di tali danni.

premetto che la tutela dell'ambiente, unitamente ad una crescita sostenibile, rappresenta la più importante delle sfide del nostro futuro; eppure, questi temi non sono ancora al centro dell'agenda politica di molti Paesi, compreso il nostro. Alla luce di quanto premesso, il provvedimento in esame desta in noi qualche perplessità: se condividiamo l'esigenza di chiarire la portata del quinto comma dell'articolo 137 del codice ambientale, ci rendiamo però conto che esso circoscrive l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui oltre a superare i valori limite previsti si scarichino specifiche sostanze, indicate nella tabella 5.

appare quanto mai necessario potenziare tutti gli strumenti di controllo al fine di salvaguardare l'integrità e la salute dei cittadini. Le ragioni sopra esposte e le perplessità descritte ci portano a dichiarare un voto di astensione da parte del Gruppo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'inquinamento idrico è causato da differenti fattori, quali gli scarichi di attività industriali o delle normali attività umane che giungono nei corpi idrici senza opportuno trattamento. È un problema che riguarda le città, quando l'acqua si riversa senza autorizzazione e senza alcun trattamento di depurazione nei fiumi o direttamente nel mare; che riguarda le industrie, e in tal caso la sua composizione varia a seconda del tipo di processo produttivo; che riguarda infine le attività agricole, per le quali va considerato l'impatto degli scarichi sul terreno e i rischi di contaminare le falde acquifere o i corpi idrici superficiali. Alcune sostanze chimiche presenti nell'acqua non trattata possono essere particolarmente tossiche: tra queste, il rame, lo zinco, il piombo, il manganese, il cromo, i solventi clorurati, gli oli minerali e gli idrocarburi. Per questo il codice ambientale, e prima ancora il decreto legislativo n. 152 del 1999 sulle acque, ha stabilito limiti e parametri, superati i quali scatta un regime sanzionatorio preciso, che deve essere puntuale ed efficace e non può essere modificato correttamente al di fuori del quadro generale. Poiché il Gruppo Italia dei Valori del Senato non condivide e non ha mai condiviso la pratica di apportare isolate modifiche alla normativa vigente con il solo ed esplicito fine di ribaltare singole sentenze della Corte di cassazione, occorre chiarire che il disegno di legge in esame non può e non deve aprire la strada ad un più ampio ventaglio di depenalizzazioni in materia ambientale. Il disegno di legge in oggetto, seppur migliorato dalla Commissione, consiste sostanzialmente nel ridurre, in materia di scarico di acque reflue, l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione ritenute più gravi, mantenendo la sola sanzione amministrativa per le rimanenti condotte che - sulla base della recente giurisprudenza e della lettura piana della legge quadro vigente - sono invece oggi ritenute meritevoli di sanzione penale. Questo modo frammentario e caotico di legiferare, tanto più se riferito ad un testo unico che dovrebbe mantenere stabilità e coerenza normativa nel tempo, genera confusione negli operatori del diritto e negli operatori del settore, esponendoli a continui cambiamenti, tanto più se questi consistono in modifiche di dettaglio su una materia oggetto di delega legislativa ancora aperta. Per affrontare il problema sollevato dal disegno di legge sarebbe stato necessario un approccio più graduale, in modo da applicare il criterio di proporzionalità alle diverse tipologie di scarico illecito, applicando il principio comunitario che esige sanzioni effettive e dissuasive. La normativa in esame riguarda prevalentemente gli scarichi industriali, dato che i privati sono di norma obbligati a riversare nella pubblica fognatura i propri scarichi domestici. L'impianto fognario deve essere autorizzato e i privati che vi immettono i loro scarichi devono rispettare la regolamentazione prevista per il suo utilizzo. Per questo la legge deve essere chiara e facilmente applicabile. Non sembra che le modifiche volute dal Governo abbiano questa capacità chiarificatrice, perché non incidono sui punti della legge vigente scritti meno bene. Siamo tutti consapevoli dell'importanza della tutela dell'ambiente in cui viviamo rispetto alle numerose minacce provenienti dalle svariate forme di inquinamento che la società moderna produce. L'effetto pratico dell'articolo unico del disegno di legge in esame sarebbe quello di sottrarre del tutto una molteplicità di forme di scarico di acque reflue alla sanzione penale, lasciandole al regime più favorevole delle sanzioni amministrative; da questo discendono gli emendamenti presentati. Nel frattempo, la situazione della depurazione delle acque e della qualità dei corpi idrici non sarà migliorata, per mancanza di investimenti. Un disegno di legge che si limita ad incidere su un solo articolo del codice ambientale non sembra uno strumento efficace né per dare certezza alle pubbliche amministrazioni, agli operatori e ai cittadini, né per combattere con forza il fenomeno dell'inquinamento dei corpi idrici in modo da dissuadere comportamenti pericolosi anche per il futuro.

facoltà. LEONI *(LNP)*. Come ampiamente discusso e convenuto fra tutti i Gruppi parlamentari in Commissione ambiente, lo scopo del disegno di legge è quello di definire un quadro di maggiore certezza giuridica per i cittadini, chiarendo la natura e l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di illecito relativo all'inquinamento da scarichi di acque reflue, di gravità sostanzialmente distinte: per scarichi reflui contenenti contenenti sostanze pericolose per la salute, o per scarichi reflui contenenti sostanze inquinanti ma meno pericolose. Pertanto, il disegno di legge non deve essere assolutamente considerato

della magistratura - che il riferimento alle sostanze pericolose della tabella 5 riguardi solo i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni e dalle Province autonome. Invece, l'intenzione del legislatore è quella di sottoporre a sanzione penale il superamento dei limiti delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, come arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, rame, e a sanzioni amministrative il superamento dei limiti della altre sostanze meno pericolose, come alluminio, bario, boro, ferro, manganese. Peraltro, le sanzioni amministrative, trattate nell'articolo 133 del codice, sono comunque alquanto pesanti (ma non costituiscono reato penale). Si tratta infatti di sanzioni che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, con un minimo di 20.000 euro in caso di inquinamento

che evita ulteriori equivoci. In pratica, visto che la norma riguarda le sanzioni penali, si definisce già dall'inizio della frase che si tratta delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del decreto legislativo n. quanto detto, il nostro Gruppo è favorevole al presente disegno di legge, come trasmesso dalla Commissione ambiente.*(Applausi

quando si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del codice ambientale e quando invece si applichino quelle penali previste dall'articolo 137.

Non si tratta di un alleggerimento di pene, ma semplicemente di precisazioni che si sono rese necessarie a seguito di alcune sentenze della suprema Corte di cassazione

il proprio voto favorevole. Vorrei però fare alcune precisazioni, la prima delle quali riguarda il testo. Il testo presentato dal Governo evidenzia un'assoluta imperizia sotto il profilo giuridico, e ciò in Commissione è stato rilevato. Ora, è vero che siamo pervenuti ad un testo su cui c'è l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in quest'Aula, tuttavia mi corre l'obbligo di precisare nuovamente come il testo presentato dal Governo sia scritto quanto meno in un pessimo italiano, e non entro nel merito delle questioni giuridiche. Per tale ragione, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un emendamento interamente sostitutivo,

per sostenere il testo che pur vedeva l'accordo di tutte le parti. Ciò va detto per precisare lo svolgimento del dibattito sul comma di un articolo Il secondo problema che voglio sollevare è di altra natura. Nella relazione illustrativa di tale provvedimento si menziona anche la delega che in questo momento è a disposizione del Ministro La delega è stata concessa in base alla legge 18 giugno 2009, su di essa il Partito Democratico ha sempre espresso forti perplessità. Capisco che questa sia una mera correzione di una piccolissima parte del codice ambientale, ma vorrei ricordare all'Aula che

cioè il decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò detto, confermo il voto favorevole del mio Gruppo, aggiungendo però che persino quando siamo d'accordo fate di tutto per emarginarci e per lasciarci nell'angolo.

il dibattito ha evidenziato la ragione principale per la quale il Governo ha proposto questo disegno di legge, ossia ripristinare la volontà legislativa degli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, in piena conformità con i principi comunitari, tra l'altro ribaditi recentemente nella nuova direttiva, prevede la proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni ambientali e anche il cosiddetto doppio binario tra sanzioni di tipo amministrativo e sanzioni di tipo penale.

una sanzione amministrativa, e circoscrivendo alla copertura del diritto penale le sanzioni più gravi. e questa necessità non ci devono però esimere dal riflettere sull'opportunità che vi sia una differenziazione e una proporzionalità di sanzioni, non solo perché voluta dal diritto comunitario, ma anche perché in alcune fattispecie la sanzione amministrativa, per le sue modalità di applicazione, è decisamente più difensiva per l'ordinamento di quanto non sia la sanzione penale. Ricordo ai colleghi che il diritto penale e le sanzioni penali si basano sulla volontarietà del comportamento, che si ricava dal dolo o dalla gravità della colpa in caso di negligenza o imperizia; invece la sanzione amministrativa opera di per sé e quindi, con multe da 20.000 euro in su, sanziona comunque il malfunzionamento di impianti o eventuali rotture che non sempre sono riconducibili ad una colpa grave o ad un comportamento doloso. Pertanto, contrariamente a quello che si può pensare, talvolta la previsione di una sanzione penale ha una efficacia di prevenzione inferiore rispetto a quella di una sanzione amministrativa. Se vogliamo fare qualche esempio, basta vedere come il codice della strada, evolvendosi nella direzione di forti sanzioni amministrative e diradando le norme penali, abbia trovato una effettività sanzionatoria ben superiore rispetto a quella che precedentemente veniva garantita.

contrariamente a quanto oggi qualche spunto polemico ha fatto apparire in Aula, è stato fortemente condiviso, fino al punto da provocare una certa rilassatezza che può aver causato l'incidente della mancanza del numero legale, forse perché qualcuno che condivideva il testo lo ha fatto valere. Non credo però si debba additare questo piccolo passaggio legislativo come una pagina di scarsa collaborazione fattiva fra le forze politiche in Commissione, o di mancata apertura del Governo rispetto ad un provvedimento che difendiamo per la sua natura e per la sua giustezza di fronte alla necessità di garantire un giusto presidio sanzionatorio dell'insieme dei comportamenti pericolosi per l'ambiente. Per tutto questo, a nome del mio Gruppo dichiaro convintamente il voto favorevole.